la costruzione di una difesa comune europea costituisce un argomento di grande attualità, che mette in evidenza la stretta connessione tra i temi della sicurezza interna ai singoli Stati membri e quelli della sicurezza a livello di Unione e a livello globale. La regione europea è più instabile e meno sicura che in passato: le crisi presenti dentro e fuori dai confini dell'Unione europea stanno impattando direttamente sulla vita dei cittadini europei, la cui richiesta di maggiore sicurezza si rinnova con sempre più forza. Le minacce da fronteggiare sono complesse nella loro natura e vaste geograficamente e nessuno degli Stati europei ha le forze e le risorse necessarie per attuare un'efficace azione di contrasto. A tal fine, appare necessario adottare un approccio flessibile e articolato anche in termini di coordinamento degli strumenti diplomatici, militari, economici, finanziari e informativi, condividendo anche le modalità e le strategie di attuazione degli stessi. La necessità di conseguire una cooperazione rafforzata e un piano comune sulla difesa europea si fa sempre più urgente. Non c'è più tempo per le incertezze e serve una risposta coordinata in grado di valorizzare in modo sinergico le potenzialità esprimibili dalle forze europee.

si può progettare una difesa comune europea quando ancora l'Europa non ha raggiunto quell'unità e quegli obiettivi previsti dai trattati istitutivi, quando ancora non si è giunti a un'Europa sociale, a un'Europa che migliora la vita dei cittadini? Come si può dare fiducia, affidare la nostra sicurezza e cedere sovranità nazionale nel difendere i nostri confini a un'Europa ancora contaminata da interessi territoriali, in cui si usa una politica di *austerity* in maniera strumentale per avvantaggiare Paesi a scapito di altri (vedi Germania)? Noi siamo un Paese non nuclearista per costituzione, ci siamo impegnati con tanto di trattato di non proliferazione nucleare a non produrre, non detenere e non utilizzare armi nucleari. Come potremmo essere coerenti con questo principio, unendoci in una difesa comune con Paesi quali Francia e Germania, che producono armi nucleari? Chi ci garantisce che non saremo obbligati anche noi ad assecondare politiche di riarmo nucleare, nell'ambito di una politica comune di difesa con altri *partner*? Come incide questa difesa comune sulle nostre leggi, i nostri valori e le nostre scelte di politica estera? Siamo già all'interno della NATO che, nonostante abbia perso la sua ragion d'essere, ci vincola portandoci in giro per il mondo a fare guerre. Inoltre, chi sarebbero i nostri *partner*? Con la Brexit anche lo scenario cambia. Perdendo Londra, l'Unione europea perde una delle due potenze militari con un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Resta la Francia - è vero - con le sue velleità nazionali e con una politica estera spesso non condivisa dai nostri *partner*, soprattutto con noi. Come funzionerebbe il processo decisionale? Rimangano sullo sfondo tanti nodi, che andrebbero sciolti subito con un dibattito parlamentare serio bisognerebbe farlo prima di manifestare a livello internazionale entusiasmi o atteggiamenti trionfalistici. Quando lo faremo? Signor Presidente, signora Ministro, la costruzione di una difesa comune europea ha mosso i primi passi a Bratislava, lo scorso settembre. L'incontro è stato un primo passo verso la concreta attuazione del piano previsto dai trattati e la strategia globale dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su come rafforzare rafforzare ovviamente la cooperazione europea in materia di difesa. Nell'ambito del processo di concreta attuazione della politica di difesa, signora Ministro, lei si accinge a presentare al Parlamento europeo una proposta italiana in merito. Le chiedo pertanto all'interno del *paper* italiano quale sia il ruolo assunto dall'Italia. Si garantisce all'Italia un ruolo chiave nella strategia di difesa del bacino del Mediterraneo, considerato anche il ruolo primario del nostro Paese nella gestione dei flussi migratori? Infine, il ritiro della Gran Bretagna dagli organismi comunitari avrà probabilmente impatti diversi sulla difesa e sicurezza europea. Quali possono essere le ripercussioni per l'Italia nell'ambito della politica di difesa comune derivanti dall'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea? Signora Ministro, vorrei sapere se il Governo non consideri l'avvistamento di due cacciabombardieri russi sui cieli della Bretagna o là vicino un atto che dimostri un grave deteriorarsi dei rapporti con la Russia; se non ritenga che questo possa essere in qualche modo una reazione alla pressione delle armi e delle esercitazioni della NATO ai confini con la Russia; se non ritenga che questa tensione da guerra fredda - scrivono i giornali - tra Europa e Russia non ci distolga dall'obiettivo comune, cioè la battaglia contro il terrorismo e l'ISIS in Siria, dove gli alleati gli alleati dei russi compiono azioni deprecabili come il bombardamento di ospedali e di civili; ma noi consideriamo laggiù alleata un'organizzazione al-Nusra che qui diciamo essere terrorista come al-Qaeda, di cui peraltro è un'affiliazione. se su tutto questo il Governo non intenda avviare un dibattito anche in Parlamento, magari con una sessione speciale sulla politica estera, visto che con tutta evidenza il quadro mondiale sta cambiando e le tensioni si moltiplicano. Signora Ministro, poiché sia la diplomazia che la Difesa italiana sembrano credere nelle prospettive della cosiddetta difesa europea, di cui si parla addirittura dall'inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso, anche se poi poco si è realizzato di concreto; poiché la divaricazione degli interessi nazionali dei principali Paesi dell'Unione europea è evidente in molti teatri, posto che la percezione della minaccia ha caratteristiche profondamente diverse da Paese a Paese; poiché è inoltre evidente che la competizione in teatri estremamente sensibili come il Mediterraneo e i Balcani, ma soprattutto - come ha illustrato il collega Mineo - è problematica ai confini della Federazione Russa, chiederei in che modo il Ministro immagini sia possibile promuovere un'effettiva integrazione europea nel campo della difesa che non privi il nostro Paese della sua sovranità militare, ma soprattutto della capacità di affermare i propri interessi anche in zone in cui non esiste un'effettiva convergenza con i *partner* del nostro Paese.

una perdita di tempo rispetto a un'Europa che rischia di implodere al proprio interno per ben altri motivi. Anche questo è segno di una crisi europea. Mi sembra, quindi, tempo perso

vari Paesi avranno le mani libere. Non so cosa ci aspetta da qui a qualche anno perché, purtroppo, se una cosa seria l'Unione europea ha fatto, è stato di impedire le solite rotture all'interno dell'Europa che hanno causato disastri e guerre mondiali. Questo è il dato reale,

stessi - che l'Italia ha il diritto di avere un esercito normale, che non dipenda da altri? Abbiamo tecnologie elevatissime, che spesso vendiamo; abbiamo uomini e intelligenze. rivedere, se possibile, il problema di avere non la cosiddetta naja, ma qualcosa in più: un esercito, certo, più numeroso, perché i tempi che paventiamo possano arrivare potrebbero essere pesantissimi.

Prepariamoci perché anche gli Stati Uniti molleranno completamente l'Europa, quindi o sapremo difendere noi i nostri confini, i nostri legittimi interessi, o saremo fuori. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le domande; ho visto che ci sono anche pareri discordanti all'interno delle domande stesse, ma credo che qui affrontiamo un tema che, al di là delle differenze di opinione, sicuramente è centrale nel dibattito che si sta svolgendo oggi in Europa. È vero, della difesa europea non ne parliamo da oggi; in realtà, subito dopo la Seconda guerra mondiale i padri fondatori dell'Europa avevano cominciato a parlare di questo tema, e sappiamo anche perché ci sono state battute d'arresto, mai per responsabilità dell'Italia, che ha sempre avuto su questo un atteggiamento europeista. Oggi, però, questo tema riprende vigore e ci sono una nuova attenzione e anche una nuova tensione da parte di diversi Stati europei per valutare la possibilità di costruire un percorso comune. Anche nella discussione di Bratislava non tutti la pensavano allo stesso modo: ci sono state Nazioni, come la Francia e la Germania, con cui l'Italia ha dialogato da da subito, molto propense a fare passi in avanti; ce ne sono state altre, come alcuni Paesi dell'Est, più preoccupate comunque che ci ci fossero fughe in avanti. Quindi, il dibattito è aperto, ma è un cantiere nel quale ritengo sarebbe sbagliatissimo non far sentire la voce italiana. Condivido in pieno l'intervento e la domanda della senatrice Amati, mentre vorrei dire al senatore Tarquinio che nessuno ha mai parlato - almeno io non l'ho mai fatto, altri sì, ma non in Italia - di esercito europeo; nessuno sta pensando di smantellare le forze armate nazionali per costruire un esercito europeo. Noi stiamo parlando di una difesa europea, che è cosa diversa: vuol dire,

si doti di una capacità sinergica di intervenire, non in contrasto con la NATO. Del resto c'è praticamente una

che ho avuto pochissimi giorni dopo la Brexit, il Ministro inglese ha inteso dire che il suo Paese intende continuare tutte le collaborazioni in atto, compresa la presenza nella missione europea EUNAVFOR Med, sulla quale vuole investire maggiormente mettendo un'altra nave.

quello è lo scenario principale in cui l'Europa dovrà muovere la propria strategia e capire i propri interventi. Di cosa concretamente si sta discutendo se non dell'esercito europeo e se non di smantellare le difese nazionali? nazionali? Già oggi la Difesa agisce sempre in modo interdipendente; noi agiamo in organizzazioni come la NATO, l'ONU e l'Unione europea ed è difficilissimo che ci siano interventi che non abbiano un consesso ampio di organizzazioni;

Il rafforzamento a livello europeo della capacità di reagire a livello operativo (perché non c'è dubbio che finora abbiamo visto molte lentezze)

L'Italia propone che a livello politico-istituzionale venga definita una vera e propria strategia per la difesa europea come piano d'implementazione degli aspetti di sicurezza e difesa contenuti nella strategia globale europea.

non c'è neppure un luogo formale in cui si incontrano i Ministri della difesa: il *forum* è una sede informale. Anche all'interno del Parlamento europeo, ad occuparsi di difesa è soltanto una sottocommissione. Quindi, è chiaro che se si vuole procedere ad un rafforzamento, anche il livello

condividendo un percorso per la formazione e l'addestramento militare comune, condividendo le forze e le capacità degli Stati membri, per giungere ad una maggiore integrazione dei nostri strumenti di azione. I Trattati europei

ciascuna Nazione europea non ha una capacità tale, nel caso in cui dovesse fare una mobilitazione molto ampia, da avere tutti i vettori aerei necessari. Firmando questo Firmando questo Trattato non abbiamo perso capacità, ma le abbiamo aumentate, perché se avremo la necessità, potremo chiedere a tutti gli altri Stati firmatari di fornirci i loro vettori e la stessa cosa possono fare gli altri Stati nei Concludendo, c'è poi tutta una parte che riguarda l'industria, su cui abbiamo presentato un *non-paper* importante, perché pensiamo che

Non avrei quindi problemi o preoccupazioni. Le nostre forze armate sono molto stimate nel mondo perché capaci, ma è certo che per le sfide che abbiamo davanti - come diceva anche la senatrice Amati - non possiamo che immaginare una risposta che sia di dimensione europea.

la Russia è fondamentale per risolvere alcune crisi, come quella siriana, che è drammatica. Detto ciò, assistiamo senza dubbio ad una *escalation*. Ciò che però abbiamo sempre fatto e continueremo a fare è provare a riportare tutti su tavoli di dialogo.

a nessuna delle mie domande: è riuscita a dribblarle in maniera incredibile. A me sembra che lei stia operando a livello europeo in un contesto in cui non le interessa la difesa in sé, ma l'industria bellica italiana.

ma mai e poi mai abbia messo i diritti dei cittadini europei davanti a tutto. Di questo me ne dispiaccio e spero che in un prossimo futuro riesca a rispondere alle domande che le ho rivolto.

Pare che in Siria si stia per fare la stessa cosa. La Russia sta tamponando e combattendo su quel fronte. Abbiamo interessi completamente diversi; per cui, ragionando di un sistema di difesa comune, è bene mettere le forze assieme, però bisogna

Signor Presidente, signora Ministro, la situazione della Libia è sempre più preoccupante, perché la gravità della crisi interessa un'area strategica per l'equilibrio del Mediterraneo e ha conseguenze molto pesanti sul flusso dei migranti in arrivo in Italia, un impegno che il nostro Paese porta anche pesantemente in Europa. Le operazioni militari avviate dalle forze del generale Khalifa Haftar nell'area della mezzaluna petrolifera, dove sorgono i principali impianti delle compagnie internazionali e italiane, rischiano di avere un effetto destabilizzante sul processo di stabilizzazione e di pace in Libia. Come è stato da lei puntualmente illustrato in Commissione difesa, oggi le nostre forze armate sono impegnate in Libia nella missione Ippocrate, finalizzata a realizzare un presidio ospedaliero in supporto alle forze libiche, così come da richiesta formale del *premier* al-Sarraj che il nostro Paese sostiene, un intervento localizzato sul territorio di Misurata. Le chiedo, quindi, un aggiornamento sullo stato di attuazione della missione e anche una conferma delle finalità della stessa. Come parlamentari del territorio cuneese, devo dirle che insieme agli onorevoli Chiara Gribaudo e Mino Taricco seguiamo con attenzione e preoccupazione anche una vicenda che interessa

Signor Presidente, signor Ministro, le chiedo se ritiene che il Parlamento italiano abbia il diritto di conoscere i limiti dell'intervento e le regole d'ingaggio del contingente militare a difesa del personale e dell'ospedale di Misurata. Inoltre, considerate la presenza dei nostri militari in Libia e la collaborazione tra i servizi dei due Paesi, non crede che il Governo si debba impegnare per ottenere le risoluzioni ONU e il consenso del Governo di Tripoli sia per avviare la seconda parte della fase 2 di EUNAVFOR Med, che prevede la possibilità

signor Ministro, schierando noi a Misurata un contingente militare nazionale che risulta al momento il maggiore contributo armato di un Paese occidentale alla stabilizzazione della Libia, l'Italia ha fatto una chiarissima scelta di campo non soltanto contro lo Stato islamico, ma anche contro le forze che sostengono il generale Haftar e quindi l'Egitto e, se vogliamo, in misura minore anche la Francia. Risulterebbero, infatti, impegnati a fianco di Tobruk contingenti di consiglieri militari sia emiratini sia egiziani. Stante che il generale Haftar recentemente si è recato a Mosca per chiedere alla Russia forniture militari, che non si sa ancora se e in che misura verranno concesse, la situazione espone sicuramente le truppe italiane al rischio di prendere parte attivamente a una guerra civile ad altissimo potenziale di internazionalizzazione. Le chiedo pertanto, signor Ministro, in che modo il Governo intenda reagire qualora le truppe al comando del generale Haftar intendano attaccare la Libia occidentale ora sotto il controllo del Governo di accordo nazionale libico.

nell'area della città libica di Misurata, rispondendo alle richieste del Governo libico per un'azione umanitaria coerente con la risoluzione ONU. In particolare, risulta che l'Italia avrebbe inviato circa 65 medici e paramedici militari, allestendo un ospedale da campo presso l'aeroporto di Misurata,

paracadutisti della Folgore. Le chiediamo, signor Ministro, se conferma la portata del contingente inviato lo scorso settembre, se tra le ipotesi per gestire la crisi libica nei prossimi mesi vi sia anche l'invio di ulteriori contingenti militari del nostro Paese, per fini umanitari o per eventuali operazioni militari, e quali proposte sono allo studio per dare una prospettiva politica genuinamente europea a futuri interventi in Libia, considerata la sostanziale disomogeneità di valutazioni e sostegni politici tra i *partner* europei in quella delicatissima zona di crisi.

esiste quasi esclusivamente nella città di Tripoli. Le milizie di Misurata sono molto infastidite dalle pretese di quel Governo e spingono per un'azione autonoma. Il generale Haftar ha conquistato il controllo dei pozzi petroliferi. Vorrei sapere se, in siffatte condizioni, non sia priva delle necessarie ragioni di sicurezza e non conveniente la nostra presenza in Libia. La prego di non rispondere dicendo che in Libia noi proteggiamo solo un ospedale, perché i giornali sono pieni di sue dichiarazioni e di dichiarazioni dell'ambasciatore americano in Italia, di generali e di osservatori che collegano di continuo questa piccola presenza alla possibilità di un intervento vero e proprio in Libia. Da qualche parte, quindi, di questo si sta parlando; in Parlamento no e soprattutto non si parla delle condizioni incredibili e pericolose della Libia nell'attuale momento.

può spiegarci in modo preciso e puntuale i passaggi autorizzativi o le votazioni che il Parlamento ha effettuato per mandare i militari italiani in Libia? Le chiedo in maniera precisa, in primo luogo, chi ha votato e quando l'invio di 40 uomini delle forze speciali nel mese di marzo in Libia; in secondo luogo, chi ha votato l'autorizzazione all'uso della base di Sigonella per gli americani per bombardare in Libia; infine, chi ha votato la famosa missione Ippocrate, che autorizza ben 300 militari ad andare in Libia. Le chiedo tutto questo come esponente del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto sono i cittadini fuori a voler sapere se l'Italia è o meno in guerra. non sono d'accordo su tutto il resto, ma su questo sì - formulo una domanda precisa. I nostri militari sono lì.

I francesi sono lì. Haftar oggi ha fatto una dichiarazione pericolosissima: ha detto che l'Italia dovrebbe lasciare l'accordo con al-Sarraj, perché loro,

essere fuori dal mondo. Vogliamo essere una Svizzera e non lo siamo, anche se la Svizzera è militarmente molto più attrezzata di noi. Il dato reale è questo. Quanto resisteremo? Questo Paese

L'8 agosto il presidente al-Sarraj ha scritto una lettera al presidente Renzi chiedendo di costituire un ospedale militare da campo.

non so se il senatore Santangelo fosse presente - sono state fatte delle votazioni con le quali non soltanto le forze di maggioranza che sostengono questo Governo, ma anche molte altre forze politiche,

dalla cosiddetta risoluzione Ruffino che regola - come sapete - le questioni che riguardano le missioni; non solo, ma anche come previsto dalla nuova legge quadro sulle missioni internazionali, che prevede questo tipo di passaggi. Queste sono le votazioni che sono state

rispondo così al senatore Mineo - opera solo nell'ambito per il quale è stato richiesto l'intervento. Nello specifico - per rispondere alle senatrici Bianconi e Manassero sarà costituito da: un'aliquota per la funzione sanitaria vera e propria, composta da 65 medici e infermieri, come lei ha ricordato; una seconda aliquota composta da 135 unità per la funzione di supporto logistico generale che servirà alla manutenzione dei mezzi e delle apparecchiature, alle comunicazioni, alla gestione amministrativa, all'organizzazione e direzione delle attività e a tutti i servizi necessari alla vita quotidiana del personale; una terza aliquota composta da 100 unità dedicata alla protezione del contingente, tanto nella fase di realizzazione dell'ospedale da campo quanto nella sua operatività. Dato che siamo consapevoli che esistono ancora molte fragilità all'interno della compagine governativa libica, come è stato ricordato in alcuni interventi, e vi è una situazione di tensione presente con il generale Haftar, insieme a questi uomini sono presenti un C-27J e una nave di Mare Sicuro, prospiciente le coste della Libia, perché, se dovessero esserci situazioni di difficoltà, ovviamente noi dobbiamo portare in sicurezza il nostro personale. Ci auguriamo che non ve ne sia bisogno. Per ora stiamo operando tranquillamente e non c'è nessuna difficoltà. Lo schieramento è stato avviato il 14 settembre mediante viaggio dall'Italia alla Libia, impiegando sia vettori navali che aerei. Il 18 settembre scorso è stata raggiunta la piena operatività della prima aliquota, con capacità chirurgiche d'urgenza e dodici posti letto; inoltre, militari italiani stanno operando nell'ospedale di Misurata a supporto degli altri medici civili per alcune specialità che non erano presenti. Ad oggi sono state fornite 165 consulenze mediche, 13 consulenze infermieristiche, 29 medicazioni chirurgiche, 40 interventi chirurgici. Fino ad oggi sono presenti complessivamente svariati medici (i numeri ve li ho già dati precedentemente). Si prevede che l'ospedale da campo raggiunga la piena operatività tra il 15 e il 20 ottobre prossimo. A quel punto saranno disponibili ulteriori capacità come: neurochirurgia, chirurgia maxillofacciale maxillofacciale e vascolare e della mano, e 50 posti letto. Passiamo invece al tema più politico. Ovviamente la necessità di una prospettiva politica europea nei confronti della Libia è quantomai auspicata dall'Italia. Voi sapete che formalmente c'è sempre stata un'unità. Quanto al riconoscimento - mi riferisco al sostegno, ma anche alla condanna di alcune azioni fatte - c'è sempre stata un'unità che ha visto il ministro Gentiloni, insieme agli altri Ministri degli esteri, sia degli Stati Uniti che dei principali Stati europei, sostenere la linea indicata dalla risoluzione delle Nazioni Unite. C'è ancora del lavoro da fare - non ce lo nascondiamo - però ci sembra che, da questo punto di vista, il quadro, ancora molto fragile e difficile,

Per quanto riguarda la domanda della senatrice Pelino, esiste un tavolo di coordinamento interministeriale per affrontare, congiuntamente con le autorità locali, le problematiche migratorie il Ministero dell'interno e anche un ufficiale di collegamento della Difesa che interloquisce con le autorità libiche (perché ovviamente, lo avete citato tutti, il tema delle partenze dei migranti e degli scafisti dalla Libia per l'Italia è un problema). Per quanto riguarda le regole di ingaggio, queste sono ovviamente finalizzate all'autodifesa del contingente, come peraltro accade normalmente in questi casi secondo le regoli vigenti anche per le missioni delle Nazioni Unite aventi finalità umanitarie.

alle votazioni ho già parlato. Sulle forze speciali volevo ricordare al senatore Santangelo che l'utilizzo di forze speciali per

tutte le richieste che lei mi ha fatto hanno previsto votazioni in Parlamento; non quello dell'uso delle basi perché è una prerogativa del Governo. *(PD)*. Ringrazio il Ministro per tutto, ma soprattutto per l'impegno che viene garantito sulla vicenda che ho rappresentato.

per affrontare in modo comune - perché la missione non è solo del nostro Paese - una situazione, che come lei ha bene detto, è estremamente fragile. Indubbiamente vanno ricercate la stabilità dell'area, la pace, la sicurezza dell'attività economica economica e dei lavoratori, ma l'importanza di questa vicenda del flusso dei migranti, che così tanto ci sta preoccupando e sul quale dobbiamo lavorare non solo dal punto di vista umanitario, ma anche in prospettiva,

mi auguro che il nostro Governo persegua questa strada. Non dobbiamo infatti dimenticare che l'Italia sente più degli altri Paesi europei il peso di quanto avviene sulle coste libiche e, quindi, questa seconda fase di EUNAVFOR Med dovrebbe essere

In Libia c'è ancora una situazione dove non tutti i Paesi europei e circostanti riconoscono unanimemente il Governo di accordo nazionale del presidente al-Sarraj.

questa operazione militare e soprattutto umanitaria. Noi riteniamo che il personale medico e paramedico militare sia tra i migliori e, quindi, in un sistema sanitario libico, dove tutto è saltato, sicuramente opereranno molto bene; a loro un grande ringraziamento perché ci rendono molto fieri. Signora Ministro, mi dispiace, ma devo dirmi insoddisfatto. So bene che per ora difendiamo solo un ospedale e che il contingente è stato inviato sulla base dei voti parlamentari sulle missioni internazionali. però, Dio non voglia, qualcuno dei nostri fosse attaccato, ci troveremmo coinvolti in un conflitto di cui, come risulta da questa risposta, non conosciamo le dimensioni reali delle forze sul campo. Ci consoliamo solo con il fatto che l'ONU ha riconosciuto il Governo di Tripoli, mentre Misurata è già un'altra cosa e Haftar ha conquistato i pozzi petroliferi. Un Paese che abbia onore di sé dovrebbe prevedere e non trovarsi poi di fronte a un'emergenza. Ripeto: Dio non voglia!

attraverso un *escamotage* che ha fatto il Governo (un emendamento della maggioranza); avete dato l'utilizzo agli americani di Sigonella attraverso le prerogative del Governo. Vi siete votati in Commissione, un affare assegnato - quindi una relazione del PD - di tutta fretta

anche i generali presenti in Libano hanno dato la stessa risposta, con tanto imbarazzo; non hanno cioè il coraggio di dire la verità. La verità è che i nostri militari non sono spesso messi in condizione di difendersi. Questo è il dato reale. Prima li ammazziamo e poi ragioniamo; sempre questa diplomazia. Vogliamo prendere una lezione? Quando questo Paese capirà che siamo stati lasciati soli rispetto a tanti temi? Quando capiremo che alcuni problemi - ce l'hanno detto in faccia - o li risolviamo noi o non ci risulta nessuno? La demagogia, il pacifismo, è tutto facile; ma i problemi restano. Bisogna avere il coraggio di essere una Nazione, se lo siamo. E ciò vuole dire tante cose; vuol dire pagare anche tanti prezzi. Queste parole non esistono più. Sudditi comunque di qualcuno o questa Italia non è capace di essere Italia? Nei limiti che le appartengono, la nostra umanità non è possibile essere nessuno. Aspettare, che cosa? Nel momento in cui veniamo travolti i guai sono solo i nostri e hanno già dimostrato di lasciarci soli. Dobbiamo saper risolvere i problemi, dobbiamo saperne pagare eventualmente i prezzi e sapere che i nostri uomini vanno difesi e hanno il diritto di difendersi, non di offendere. Dobbiamo capirlo; se questa consapevolezza non c'è, povera Italia!

nell'Aula del Senato avrà luogo la commemorazione solenne, alla presenza del Presidente della Repubblica, del senatore a vita, Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. La seduta è tolta